Mentre si avvicina il Natale, in un'agonia che non finisce, Antonio Schiavone, Roberto Scola...

correttezza del loro operato, ma quanto era stato segnalato per tempo non è stato tenuto nella debita considerazione e tutto ciò è sotto gli occhi di tutti;

perché avendo presieduto quel Consiglio dei ministri avrebbe dovuto intervenire in maniera corretta. Non vorrei però che la corsa ai ripari che è stata evocata significasse

che un ramo del Parlamento non affronti un problema tanto grave e aperto alle porte del nostro Paese.

costringeva a lavorare. Voglio sottolineare che nel 2005 un incendio virulento durato tre giorni non ha provocato morti per pura fortuna. Mi pare che la vicenda di Torino, questa disgrazia, questo omicidio di sei - per ora - operai interroghi i tempi della politica, la nostra capacità di intervenire sui fatti. C'è un aspetto importante

incentivati, moltiplicati e possano avere effetti concreti. La prescrizione deve essere misurata nel suo tempo di attuazione, altrimenti è a rischio; uno stabilimento non può funzionare se sulle condizioni pendono 30-35 prescrizioni che non vengono soddisfatte: vuol dire lasciare gli operai in condizioni di rischio assoluto. Credo che dobbiamo muoverci perché, com'è stato richiesto, i decreti attuativi siano approvati rapidamente e si operi per

che nella sola giornata di ieri ci sono state altre morti sul lavoro ed esattamente a Ceccano, Udine, Brescia, Avellino e Valenza. Altri cinque operai - sempre operai sono deceduti sul luogo di lavoro. Io non penso si tratti di morti bianche: in molti casi si tratta di veri e propri omicidi preterintenzionali. *(Applausi che la magistratura indaghi a fondo, perché rendere onore e giustizia a quei morti e alle loro famiglie significa anche far pagare i colpevoli e i responsabili di questi omicidi. Siamo vicini alle famiglie, il Senato della Repubblica è stato già ieri vicino a queste famiglie e continuerà ad esserlo in questa triste vicenda. **Sui

che lancia un segnale forte di attenzione da parte del Governo e della maggioranza al comparto agroalimentare, che rappresenta uno dei settori di punta della nostra produzione nazionale.

alla Francia. Il settore agroalimentare, tra l'altro, recentemente - tre anni fa - ha superato quello tessile nella graduatoria dei settori industriali più sviluppati nel nostro Paese, raggiungendo il secondo posto dopo l'industria metalmeccanica. Si tratta di un comparto sicuramente importante per l'economia nazionale; soprattutto, si tratta di un comparto importantissimo per la vocazione esportatrice della nostra Nazione. Il *made in Italy* agroalimentare è apprezzato conosciuto in tutto il mondo; non a caso viene imitato con la cosiddetta agropirateria. Abbiamo coniato questo neologismo per definire

nella sola, grande distribuzione statunitense soltanto l'8 per cento di quello che viene ricondotto al *made in Italy* *sounding* è realmente prodotto in Italia; tutto il resto (più del 90 per cento) l'Italia non l'ha vista neanche in cartolina. Quindi, si tratta di uno spazio di mercato nella globalizzazione dell'economia sicuramente molto rilevante, che l'Italia deve poter, invece, cogliere con la sola propria produzione. Quindi, è un settore sul quale ritengo che l'Italia debba puntare ancora di più per mantenere le proprie quote di mercato a livello internazionale. internazionale. La manovra di bilancio in agricoltura si distribuisce sui tre provvedimenti che hanno caratterizzato la manovra finanziaria di quest'anno. Mi riferisco alla legge finanziaria, al decreto fiscale

Il problema dei controlli per combattere l'agropirateria e le contraffazioni delle produzioni nazionali ad opera dei nostri concorrenti esteri è uno dei temi che anche in quest'Aula, è soprattutto in Commissione agricoltura, abbiamo dibattuto spesso.

importante problema, quello cioè della garanzia della sicurezza alimentare per i nostri consumatori. Da un lato, quindi, si tratta di difendere i nostri prodotti tipici dalle contraffazioni, dall'altro, si tratta di garantire ai consumatori italiani la sicurezza alimentare. Ecco allora che in finanziaria sono stati stanziati 25 milioni di euro per l'attività specifica di Agecontrol Spa, finalizzata proprio alla lotta alla contrattazione e alla

per passare poi all'imposta di registro ridotta per l'accorpamento della proprietà coltivatrice, fino ad arrivare alle agevolazioni fiscali alla pesca e all'accisa zero per il gasolio impiegato nelle serre.

contiene una sorta di interpretazione autentica di varie norme prima sparse in diversi provvedimenti, anche con alcune contraddizioni interne.

anch'essa nel decreto sul *welfare*, riguarda la possibilità per le imprese agricole di accedere alla cassa integrazione straordinaria, che fino ad oggi era stata negata e che rappresenta una grande innovazione rispetto al passato. Ci sono poi incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e norme importanti per la sicurezza sul lavoro, di cui abbiamo appena parlato all'inizio di seduta, poiché è uno dei temi di maggior gravità

intensificano la lotta agli incidenti sul lavoro a garanzia della sicurezza sul lavoro. Ci sono poi norme sul finanziamento alla formazione, sul riordino degli interventi a favore dell'occupazione nelle imprese colpite da calamità naturali. Inoltre, chiudendo la parte relativa al lavoro, il testo contiene una importante norma di attuazione delle disposizioni relative al lavoro occasionale di tipo accessorio. Il sistema cosiddetto dei *voucher* adesso riguarda solo la raccolta dell'uva, cioè la vendemmia, ma in futuro potrà essere esteso anche ad altri lavori stagionali di raccolta agricola. Esso permette di coprire dal punto di vista contributivo e assicurativo i lavoratori impiegati in queste operazioni di raccolta con una grande facilitazione in termini di adempimenti burocratici e di comunicazione; inoltre, consentirà di regolarizzare quelle forme di lavoro, svolte magari da parenti ed amici per le fasi di vendemmia, che fino ad oggi erano completamente affidate al lavoro nero.

Innanzitutto, abbiamo chiarito la possibilità di utilizzare l'IRAP agevolata prevista per il settore agricolo anche per le cooperative forestali.

Ci sono norme sui gruppi di acquisto solidale (GAS), una forma di commercializzazione della cosiddetta filiera corta, cioè di avvicinamento fra produttore agricolo e consumatore in termini di vendita dei propri prodotti che fino ad ora non avevano trovato una sistematizzazione fiscale. I gruppi di acquisto solidale non erano previsti dalla nostra normativa fiscale e finalmente

Ci sono poi importanti norme per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato, con la previsione di nuove assunzioni per la lotta agli incendi boschivi,

unità in deroga alla normativa vigente; pertanto finalmente potremo dotare il Corpo forestale delle risorse umane necessarie per svolgere un'azione di lotta agli incendi boschivi efficace ed efficiente.

rilancia il piano irriguo nazionale anche per il decennio successivo, quindi dal 2011 in poi. Si prevede una riserva di fondi di 100 milioni annui, con contributi pluriennali quindicennali. La

Torno, quindi, alla mia premessa ribadendo che l'agricoltura agroalimentare è uno dei pochi settori su cui l'Italia può puntare per ampliare la propria quota di mercato internazionale. Su questo versante i dati dell'anno scorso attestano che le esportazioni di prodotti agroalimentari italiani hanno sperimentando un incremento molto significativo, che testimonia

non opportuna perché sicuramente si deve andare verso un riordino e, in molti casi, anche verso un accorpamento dei diversi consorzi di bonifica, ma la soppressione di questi istituti

moralmente irresponsabile perché usa la spesa pubblica, e quindi le risorse dei cittadini italiani, per tenere insieme una maggioranza che non esiste nel Paese e che nel Parlamento sta insieme senza un progetto politico alto finalizzato agli interessi degli italiani, ma pagando una lista della spesa - che si allunga ogni giorno - del particolare, del localismo egoista e miope. È politicamente sbagliato perché ritiene di usare la spesa pubblica per cercare di risolvere problemi del Paese

Il 28 settembre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato un testo con 97 articoli; il 17 novembre scorso il Senato ha votato un testo con 151 articoli e ora, dalla Camera dei deputati, è tornato un testo con oltre 1.000 commi che disegnano un provvedimento legislativamente mostruoso, che perde completamente la fisionomia di manovra correttiva di bilancio e diventa un contenitore pieno di provvedimenti destrutturati ed informi, somma di interessi locali e corporativi, di segnali politici per gratificare il proprio specifico segmento elettorale

a parte la completa inaffidabilità delle cifre riportate per le coperture, trovate ai più disparati provvedimenti di spesa, questo provvedimento aveva una dimensione economica - se ben ricordate - di 10,7 miliardi di euro quando è stato approvato dal Governo;

Vi sono riduzioni di spesa non realizzabili, a nostro avviso, o comunque sovradimensionate che si tradurranno, quando vi sarà il riscontro della gestione nell'anno a venire, in necessità di nuove tasse. Ci sono sovrastime nelle entrate a pressione fiscale invariata che, con il ciclo economico al quale stiamo assistendo a livello internazionale, certamente non potranno essere attuate. un atteggiamento criticabile se riscontrato nei bilanci di qualche Comune poco responsabile, che abitualmente tende a sovrastimare le entrate e a sottostimare le spese per far quadrare i conti di anno in anno, ma direi che è inaccettabile se riscontrato nella manovra finanziaria di uno Stato. Peraltro, l'atteggiamento da amministratore locale, anziché da legislatore nazionale che ha una visione strategica della funzionalità organica dello Stato nelle sue varie articolazioni, è evidenziato nelle decine e decine di fondi istituiti presso i vari Ministeri, che si prefiggono di agire direttamente nei più disparati settori, ignorando le leggi vigenti e saltando le competenze dei diversi enti territoriali.

sapete, in Parlamento è in corso la discussione sul disegno di legge per il governo del territorio), si stabilisce il principio della compensazione urbanistica, ovvero aree verdi in cambio di opere pubbliche. Un principio interessante, ma delicato da gestire, che dovrebbe essere inserito in una legge organica, appunto il disegno di legge in discussione, e non si comprende per quale motivo debba essere inserito in finanziaria.

nonché il numero stesso dei componenti degli organi rappresentativi, con l'evidente risultato che, ammesso che le Regioni riescano in pochi mesi a mettere in piedi ed approvare leggi con questo obiettivo, avremo una destrutturazione complessiva del sistema delle autonomie locali per quanto riguarda le comunità montane a livello nazionale e i cittadini italiani, a seconda della Regione nella quale si trovano, saranno inseriti in comunità montane oppure no, con vantaggi o svantaggi a seconda del luogo dove vivono e risiedono. Ogni Regione avrà quindi comunità montane definite su basi diverse e i cittadini, come dicevo prima, avranno vantaggi o svantaggi a seconda della parte del territorio nella quale vivono. Senato, sempre ricordando che è in corso il tentativo di scrivere il codice delle autonomie, si è voluto insistere nel ridefinire una serie di norme con l'obiettivo di ridurre le spese degli enti locali. Segnalo che in qualche caso esse aumentano, ad esempio nel caso della disposizione in cui si definisce che il presidente e gli assessori delle unioni dei Comuni, dei consorzi tra enti locali e delle comunità montane,

o del consorzio dei Comuni, evidentemente aumentando il valore dell'emolumento. Forse qualcuno non se n'è accorto, ma questo va esattamente con l'articolo 1, comma 166, si sposta nuovamente di un anno l'obbligo di passaggio da tassa a tariffa, in questo modo umiliando quelle amministrazioni comunali che correttamente avevano rispettato i termini e quindi creando, come sempre, la sensazione netta che in Italia convenga sempre fare i furbi e non rispettare le leggi, perché tanto arriva una proroga. All'articolo 2, comma 8, viene stabilito che i Comuni possono inserire nei propri bilanci di parte corrente il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione fino al 2010: è un altro segnale di abbassamento del livello di serietà delle amministrazioni comunali, che possono utilizzare fondi, che invece dovrebbero essere naturalmente indirizzati ad infrastrutturare un territorio in espansione, alla gestione di spese correnti. Passo ad alcune brevi segnalazioni sul tema dell'ambiente. È di questi giorni la pubblicazione della relazione annuale dell'ANPA, da cui emerge la situazione - che tutti conoscono - di forte criticità ambientale in alcune parti del Paese, soprattutto al Nord, nello specifico della Pianura padana. Lì abbiamo

per rendere impossibile la realizzazione di una rete moderna ed efficiente di treni, collegata al sistema europeo, per favorire il passaggio di percentuali importanti di merci dalla gomma al ferro. Dovremmo costruire centrali nucleari, per avere energia pulita, in modo da poter trasformare gli impianti di riscaldamento e teleriscaldamento ad energia elettrica prodotta a basso impatto ambientale.

per il reticolo idrografico e i versanti, gestite direttamente dal Ministero, su richiesta dei Comuni e comunità montane. Dove finisce il lavoro fatto dalle Regioni e dalla Provincia sul territorio?

che vi sarebbe una responsabilità degli uffici del Senato e, specificamente, degli uffici della Commissione giustizia del Senato. Ciò è totalmente falso. Colgo, anzi, l'occasione per dire che la politica deve smettere di scaricare sui tecnici le proprie responsabilità:

poiché poco prima su un voto di fiducia una parlamentare della maggioranza aveva votato contro e vi era il timore che il decreto potesse essere respinto. Trasmesso il provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento, e rilevatasi correttamente la necessità di modificare quella norma, dei deputati la via maestra di emendarla, e ciò non per responsabilità di qualche tecnico ma per la preoccupazione, tutta politica, che se il decreto fosse tornato al Senato in terza lettura ci sarebbe potuto essere qualche altro incidente politico. L'altra possibilità a disposizione era quella di approvare comunque il provvedimento così com'era e di affidarlo poi al presumibile intervento del Presidente della Repubblica (con lo strumento che la Costituzione gli mette a disposizione, il messaggio presidenziale,

La prima riflessione è che qualcuno sapeva in qualche modo che tale emendamento non era corretto formalmente e quindi passibile di inammissibilità. È sfuggito alla Presidenza quanto era stato detto, ma c'è una connivenza politica sul fatto che tale emendamento, assolutamente infondato, assolutamente inammissibile, è stato lasciato passare per motivi politici. Questa è la prima riflessione. Seconda riflessione. Non voglio mettere il dito nella piaga in casa di altri, ma è stata fatta un'evidente dichiarazione di imbarazzo politico all'interno della maggioranza. Ne prendiamo atto, non abbiamo bisogno di mettere in piazza più di tanto, ma ricordo a quest'Aula che un Ministro della Repubblica aveva minacciato pubblicamente le proprie dimissioni e in qualche modo esposto il proprio onore e che, a tutt'oggi, non abbiamo una risposta conseguente.

Ma ciò che oggi veramente fa male al cuore di chi ama la politica e il Parlamento è l'aver visto che un Ministro, che è poi il Ministro della giustizia (mi dispiace dirlo, perché è anche un mio vecchio amico) abbia potuto affermare: «Io con questo ho calmato i cattolici». Ma un'Assemblea parlamentare è un'Assemblea laica, nella quale ci sono cattolici, non cattolici ed acattolici: ci sono tutti coloro che, che, in funzione della propria soggettività, vengono eletti o scelti, come spesso oggi accade, dai partiti per fare i parlamentari. si può stabilire che il Ministro della giustizia (che credo dovrebbe avere doti tecniche per accorgersi che un trapianto qualche volta crea problemi di rigetto, come si è visto questa volta)

proposta. Infatti, la legge qui nasce, ma poi vola per conto suo e va verso la collettività, sfiorando i tetti di tutte le case, dove vi sono uomini e donne di buona volontà che dovrebbero sperare che la legge,

Ci può essere il dolo, ci può essere la colpa, ci può essere la disattenzione, ma aver detto da parte di un Ministro che si fregia del titolo non più, per fortuna, «di grazia», ma di giustizia che la questione veniva stabilita in relazione alla cattura di voti eventualmente renitenti dei cattolici è una cosa così grave, signor Presidente, che può essere scritta sui titoli dei giornali senza che nessuno si indigni, ma rispetto alla quale, se un parlamentare si alza e dice che queste cose così non si fanno, Diceva il professor Biondi, che si chiamava come me ma era un cultore del diritto romano, in dialetto toscano: «E 'n si pole e 'n si deve», cioè non si può e non si deve stabilire un rapporto in cui l'emendamento si inserisce surrettiziamente, si dice che poi lo si toglierà si cattura così un voto di fiducia magari di un senatore a vita venuto, come ha fatto l'altro giorno il senatore Cossiga, ad arricchire di *calembours* un discorso in cui la coerenza non era la regina dell'opinione e nemmeno della decisione.

autorevole esponente politico apparse su importanti giornali, inaccettabili perché i fatti non sono questi ed ora il presidente Salvi con onestà intellettuale li ricostruisce. Voglio ricordare come prima il presidente Buttiglione e poi il presidente Pera avevano detto con chiarezza che c'era un errore. Il fatto che non si sia inteso correggerlo e si sia andati avanti con quei comportamenti del ministro Mastella che testé il senatore Biondi ricordava ci dice che veramente c'è non solo disorientamento all'interno della maggioranza, non solo incapacità, ma c'è un'impossibilità di agire in modo chiaro, lineare, corretto, serio e ciò è dovuto ai contrasti enormi che questa maggioranza ha al suo interno. Dunque noi, ribadendo ancora una volta che queste cose non devono succedere, che intendiamo denunciarle con forza, auspichiamo che questa maggioranza ponga fine alla sua azione, così non si può andare avanti: qui c'è un interesse del Paese che è diverso dall'interesse di questa maggioranza ed è evidente che deve prevalere l'interesse del Paese. finestra"). Passiamo alla discussione del Documento IV-*bis*, n. 3, recante: «Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di ministro della giustizia *pro tempore*, nonché dei signori Marco Preioni, Fausto De Santis, Daniela Bianchini, Alfonso Papa e Giuseppe Magni,

La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari propone all'Assemblea il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Roberto Castelli nonché degli altri soggetti. L'Assemblea delibererà separatamente su ciascuna di tali proposte di diniego. Tali proposte, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo 135-*bis* del Regolamento, s'intenderanno respinte qualora non conseguano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, cioè 162 voti. Nella seduta di oggi esauriremo la fase della discussione. Le votazioni avranno invece luogo nella seduta antimeridiana di domani, dopo le due votazioni finali su bilancio e finanziaria, con la facoltà - per coloro che non abbiano preso parte alle votazioni elettroniche - di dichiarare il voto ai senatori segretari fino alle ore 19 di domani. Avverto che, dopo l'eventuale intervento del relatore, senatore Manzione, potrà intervenire un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti. Chiedo al relatore, senatore Manzione, se intende integrare la relazione scritta. onorevoli colleghi, il 24 novembre 2006 il Collegio per i reati ministeriali presso il tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Castelli, nella sua qualità di ministro della giustizia *pro tempore*, nonché di altri indagati (Marco Preioni, Fausto De Santis, Daniela Bianchini, Alfonso Papa e Giuseppe Magni)

Il procedimento, trasmesso alla Giunta per le determinazioni di competenza e poi all'Aula, costituisce uno stralcio di un più vasto procedimento penale. Tra il 2001 e il 2003, il ministro Castelli con propri decreti conferiva a Giuseppe Magni un incarico avente ad oggetto i problemi dell'amministrazione penitenziaria in genere, e quelli dell'edilizia penitenziaria in particolare, valutati anche in relazione ai rapporti con altri Ministeri. Tra il 2002 e il 2003, il ministro Castelli conferiva poi con propri decreti a Gian Mario Airoldi un incarico avente ad oggetto i problemi dell'edilizia giudiziaria, con particolare riguardo ai rapporti con gli enti locali. Infine, il Collegio per i reati ministeriali ha preso in esame altri due incarichi di durata semestrale conferiti, sempre dal ministro Castelli con propri decreti fra il 2001 e il 2002, ad Amedeo Maffei, aventi ad oggetto il supporto psicologico degli operatori carcerari e l'analisi dei problemi psicologici dei detenuti. In data 17 maggio 2007, il dottor Marco Preioni, il dottor Fausto De Santis, il dottor Alfonso Papa e la dottoressa Bianchini - tutti coindagati e componenti del comitato di valutazione - hanno depositato una propria memoria, con la quale si richiamava innanzitutto l'attenzione sul fatto che il conferimento di incarichi a consulenti esterni corrispondeva ad una prassi consolidata, di cui si erano avvalsi già in precedenza altri Ministri della giustizia a cominciare dal ministro Flick, e che le carenze organizzative del sistema di articolazione della struttura del Ministero della giustizia, all'epoca dei fatti, risultavano evidenti. Erano infatti sempre maggiori e molteplici le competenze facenti capo al Ministro quale organo di indirizzo politico, per l'espletamento delle quali non poteva obiettivamente farsi riferimento alle strutture ministeriali, in particolare alle varie direzioni generali ed ai magistrati addetti alle stesse, poiché funzionalmente inidonei a farsi espressione di un rapporto fiduciario tipico di una funzione di indirizzo eminentemente politico. In conclusione, la memoria dei coindagati rilevava che i membri dei comitati, tutti dirigenti o magistrati presso il Ministero, non percepivano alcun particolare compenso per l'attività di valutazione delle consulenze, svolta, quindi, al di fuori delle loro proprie competenze ordinarie. La Giunta, onorevoli colleghi, ha avuto già modo di occuparsi di recente delle problematiche concernenti il conferimento di consulenze da parte di Ministri con particolare riferimento, tra l'altro, proprio al Ministero della giustizia, in occasione dell'esame del documento IV-*bis*, n. 2, della presente legislatura, avente ad oggetto anch'esso una domanda di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione nei confronti del senatore Roberto Castelli. Nella relazione di cui al già citato documento IV-*bis*, n. 2-A, con la quale questo stesso relatore propose all'Assemblea del Senato il diniego della concessione dell'autorizzazione a procedere (relazione le cui conclusioni vennero approvate a larghissima maggioranza nella seduta del 14 febbraio 2007 da questa stessa Aula del Senato), la Giunta ritenne che fosse possibile fare rinvio al decreto di archiviazione adottato in data 13 luglio 2006 dal medesimo Collegio per i reati ministeriali per avere un'idea della situazione esistente presso il Ministero della giustizia, dal punto di vista dell'adeguatezza dell'articolazione organizzativa e della dotazione di personale di tale Ministero, nel periodo specificamente considerato. In particolare, il citato decreto di archiviazione rilevava che: «Quanto al merito della vicenda (...) è emerso che il conferimento di siffatti incarichi a consulenti esterni era ormai frutto di una prassi consolidata di cui si erano avvalsi già in precedenza altri altri Ministri della giustizia, prima fra tutti il ministro Flick (...)». Il provvedimento del cosiddetto tribunale per i Ministri proseguiva evidenziando che: «Le carenze organizzative del sistema di articolazione della struttura ministeriale risultavano all'epoca dei fatti assolutamente evidenti, in particolare con riferimento all'attività di raccordo tra il Ministro e il Parlamento (...). Analoghe carenze (...) erano ancora riscontrabili con riferimento ad altre figure professionali, alcune strettamente correlate alla funzione di indirizzo politico propria del Ministro

del Ministero della giustizia in quel momento. Il provvedimento conclude con un'affermazione: «Vi era, concludendo sul punto, una situazione di *deficit* tra le esigenze politico-amministrative da fronteggiare e la dotazione di personale a disposizione di Ministri». I rilievi che ho esposto rendono pertanto evidente come, nel periodo interessato (1999-2002), la dotazione di personale del Ministero delle giustizia risultava carente anche rispetto allo svolgimento di competenze tipiche di tale Dicastero. Tale affermazione, corre l'obbligo di ripeterlo, non è della Giunta, ma riproduce le affermazioni che lo stesso Collegio per i reati ministeriali, nell'archiviare altre posizioni in quel più complesso procedimento penale, in qualche modo rappresentava. Ora, sia dagli atti trasmessi, sia dalle audizioni svolte, appare evidente che, nell'assumere la responsabilità del Dicastero della giustizia, il senatore Castelli ha scelto di perseguire un miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa dello stesso, anche mediante l'apporto di contributi ed esperienze provenienti dal mondo dell'impresa e da quello delle realtà amministrative locali. È innegabile che ci si trova di fronte ad un approccio sostanzialmente coincidente - dal punto di vista metodologico - con quello che, ad esempio, il ministro Flick nella XIII legislatura aveva messo in campo, cioè con la volontà del titolare della funzione di indirizzo politico di perseguire un miglioramento dell'efficienza dell'apparato ministeriale, mediante il contributo di esperienze provenienti da contesti diversi (per il ministro Flick si trattava del contesto e dell'ambito accademico; per il ministro Castelli del mondo dell'impresa e delle amministrazioni locali). Ad avviso di questo relatore che, occorre ribadirlo, ma risulta dagli atti, non è stato mai tenero nei confronti dell'ex ministro Roberto Castelli, non è compito né della Giunta né dell'Assemblea del Senato formulare un giudizio politico circa la condivisibilità ovvero l'opportunità delle diverse impostazioni sopra indicate, posto che nessuna di esse appare manifestamente irragionevole. Ciò che invece appare indubbio - e rilevante ai fini delle determinazioni di competenza, prima della Giunta e adesso dell'Assemblea - è che la scelta fatta dal senatore Castelli nella sua qualità di Ministro della giustizia *pro tempore* (così come quelle analoghe dei suoi predecessori) rientra, senz'altro, fra le prerogative del Ministro in quanto titolare della funzione di indirizzo politico, in relazione alle funzioni amministrative attribuite al Dicastero della cui responsabilità era stato investito. Il rilievo di un'eventuale afferenza degli incarichi di consulenza all'attività di collaborazione nell'espletamento della funzione di indirizzo politico è peraltro ammesso dallo stesso Collegio per i reati ministeriali che, a pagina 15 della domanda di autorizzazione, pacificamente ammette che, ove tale afferenza sussistesse, si tratterebbe di una «circostanza che escluderebbe ogni possibilità di sindacato in questa sede». Il Collegio per i reati ministeriali ritiene, però, che le attività svolte dai consulenti, nei casi considerati, non possano essere ritenute attinenti all'attività di collaborazione alla funzione di indirizzo politico del Ministro. Questa affermazione, però, appare smentita, ad avviso non solo del relatore ma di tutta la Giunta, o meglio della maggioranza della Giunta che ha votato la proposta formulata in Aula, oltre che dalle precedenti diverse decisioni del Collegio per i reati ministeriali, che ha proceduto ad archiviare moltissime posizioni simili riguardanti altri Ministri, anche dalle stesse risultanze degli atti trasmessi e da quanto emerso in sede di audizione. audizione. Se la caratteristica specifica e quindi l'impronta politica che il ministro Castelli ha dichiarato fin dall'inizio di dare alla sua attività politica è stata quella di recuperare efficienza, e tutto questo

che comunque va fatto un ragionamento preliminare. In termini generali, è necessario precisare fin d'ora che, per la Giunta, le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, conformemente a quella che sembrerebbe la lettura più corretta dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ricomprendono non solo la definizione di obiettivi, priorità, piani, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione, ma anche la verifica della rispondenza dei risultati dell'attività e della gestione agli indirizzi impartiti. In un simile quadro, rientra quindi in modo del tutto fisiologico sia l'attività di persone di fiducia del Ministro, che seguono specifiche aree del Dicastero di competenza e che a lui riferiscono sulla situazione di fatto esistente, sia le attività volte alla realizzazione di progetti innovativi, che possono poi essere utilizzati come modello per la definizione in futuro di nuovi programmi di azione politico-amministrativa. Sulla base di tale definizione delle funzioni di indirizzo politico definizione che si rifà, come ho detto, all'articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 - la Giunta è dell'avviso che ad essa possano senz'altro essere ricondotte le attività svolte dai consulenti nei casi in esame e che, ai fini delle determinazioni di competenza della Giunta, e conseguentemente dell'Assemblea del Senato, tale circostanza sarebbe di per sé sufficiente per concludere che le condotte degli indagati sono funzionali al perseguimento di un interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo, secondo modalità pienamente conformi al quadro normativo di riferimento. La Giunta però ha preferito approfondire l'esame della situazione, proprio per avere altri elementi. In questa prospettiva, va sottolineato anche il rilievo di alcune circostanze ulteriori emerse, relative alle gravi difficoltà che il ministro Castelli dovette affrontare nel momento in cui ha assunto la titolarità del Dicastero della giustizia. In proposito, appare utile fare specifico riferimento alle dichiarazioni rese il 4 luglio 2005 dal dottor Settembrino Nebbioso, capo di gabinetto del Ministro della giustizia: «Quando parlo di una struttura disastrata, parlo di una struttura che andava creata, nel senso che c'erano ad esempio le direzioni generali, ma le direzioni generali erano state cancellate, non dovevano più funzionare, per cui bisognava creare i dipartimenti, quindi tutta una serie di provvedimenti anche nuovi da adottarsi, sui quali non si poteva fare riferimento a dei precedenti». È appena il caso di sottolineare che le dichiarazioni del dottor Nebbioso confermano in modo pieno e completo quanto affermato dal senatore Castelli, circa la situazione di estrema difficoltà in cui versava il Ministero della giustizia nei mesi iniziali della XIV legislatura, e quanto ammesso anche nella relazione del Collegio per i reati ministeriali. Passo adesso - ed è l'ultimo aspetto che tratterò, per il resto rinvio alla relazione corposa che è stata depositata - ad esaminare specificamente le singole collaborazioni. riguarda quella del dottor Magni, dagli atti emerge che egli ha svolto la sua attività in modo effettivo, contribuendo alla realizzazione di risultati che non possono essere negati come dato oggettivo e sui quali - per quanto consta alla Giunta - non risultano essere state espresse valutazioni negative nelle competenti sedi istituzionali. A titolo puramente esemplificativo, e senza nessuna pretesa di esaustività, è sufficiente considerare il contributo all'apertura del carcere di Bollate, il riammodernamento della colonia penale di Is Arenas Is Arenas in Sardegna, il lavoro svolto per la riqualificazione dell'Isola di Pianosa, la sistemazione del carcere di Arghillà, la pianificazione completa dei siti dove costruire nuove carceri, nonché il contributo alla realizzazione di un progetto di lavoro per detenuti riguardante il ricondizionamento di materiale informatico di un progetto di lavoro per detenuti relativo al disassemblaggio di materiale elettrico. In questa prospettiva appare significativo quanto affermato dal dottor Tinebra, nella sua qualità penitenziaria (DAP), il quale evidenzia che l'attività dei consulenti Giuseppe Magni ed Amedeo Maffei è stata svolta in stretta collaborazione con le articolazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, pur trattandosi in ogni caso di specifiche iniziative del Ministro, connesse alla sua attività di indirizzo generale. In particolare, per quanto riguarda il Magni, la nota, da un lato, consente di confutare l'accusa in merito ad un asserito inadempimento dell'incarico da parte del consulente (così come emerge in qualche verso nella richiesta del tribunale per i Ministri) e, dall'altro, conferma l'esistenza fra il Magni e il Ministro di un rapporto altamente fiduciario e personale. Per quanto riguarda poi le ulteriori contestazioni relative alle trasferte all'estero effettuate dal dottor Magni, per quel che concerne la trasferta in America settentrionale risulta che la stessa ha avuto ad oggetto la visita di strutture penitenziarie e incontri istituzionali sempre in materia penitenziaria; tuttavia, anche per le altre trasferte, da quella in Albania a quella a Mosca, risulta agli atti una specifica e pacifica documentazione che non illustro perché è stata oggetto, in maniera esaustiva, di una valutazione nella relazione. Quanto alla collaborazione dell'Airoldi, valgono nei suoi confronti considerazioni non dissimili da quelle svolte relativamente al dottor Magni. I risultati conseguiti dal dottor Airoldi sembrano confermare la validità e la ragionevolezza della scelta fatta dal Ministro della giustizia *pro tempore*. Dalla documentazione esaminata emerge infatti che, nel periodo in cui si è concentrata l'attività dell'Airoldi, si sia avuto un incremento significativo del volume di finanziamenti erogati tramite la Cassa depositi e prestiti per le finalità in questione. Un simile risultato, sulla base degli atti, non sembra possa avere altra spiegazione che quella fornita dallo stesso Airoldi circa l'attività da lui svolta al fine di ottenere una effettiva o diversa utilizzazione di stanziamenti che risultavano bloccati per disfunzioni amministrative locali o mancanza di un adeguato raccordo fra livello locale e livello centrale. locale e livello centrale. Questo significa che il dottor Airoldi si è fatto carico di verificare quali fossero i finanziamenti che erano stati precedentemente accordati, ma non erano stati utilizzati; infatti che quando si parla di edilizia giudiziaria intervengono direttamente i Comuni per sopperire alle esigenze dei vari tribunali; pertanto, quando tali finanziamenti non venivano utilizzati, di fatto risultavano impegnati anche se non si procedeva a realizzare il lavoro o l'attività per la quale erano stati previsti. Il dottor Airoldi ha fatto qualcosa che risulta agli atti della Giunta e che non avrebbe fatto nessun funzionario del Ministero: contattare direttamente i singoli responsabili delle amministrazioni locali, verificare se il finanziamento per quella specifica attività era ancora necessario e, qualora non risultasse necessario, fare in modo che si rinunciasse a quell'intervento per far confluire su altre attività quei fondi specifici. Quanto alla collaborazione del dottor Maffei va sottolineato come dagli atti trasmessi risultino, anche in questo caso, non solo l'effettività dell'impegno svolto dal medesimo nell'espletamento degli incarichi affidatigli, ma altresì la rilevanza quantomeno di alcuni risultati conseguiti. Valga ad esempio la nota del Provveditorato regionale per la Lombardia del 17 novembre 2003 con cui viene comunicato al medesimo dottor Maffei «del grande riconoscimento ottenuto dal progetto, a cui lei ha contribuito con peso rilevante, relativo al carcere di Bollate da parte della Cisco System International USA». Nella stessa nota si parla del progetto in questione come di un progetto unico - mediante il quale sono stati ottenuti dai partecipanti allo stesso «eccellenti risultati umani e professionali» - e suscettibile di aprire «una svolta nella concezione della riabilitazione detentiva».

le concrete modalità di svolgimento degli incarichi contestati sembrano confermare innanzitutto il loro collegamento con le funzioni di indirizzo politico del Ministro come in precedenza definite. Sulla base di quanto esposto può considerarsi altresì accertato che le consulenze in questione sono state conferite a persone in grado di fornire comunque un apporto professionale specifico e che la loro attività ha prodotto risultati concreti che nella maggior parte dei casi sono da ritenersi anche apprezzabili dal punto di vista qualitativo. Per tutte queste ragioni, la Giunta propone all'Assemblea, ricorrendo una delle due circostanze esimenti previste dall'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale n. 1 del 1989 (cioè

Signor Presidente, onorevoli colleghi, è mio compito segnalare ed esplicitare le ragioni per cui, all'interno della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, i senatori del centro-sinistra presenti al momento della votazione, fatta eccezione per il senatore Manzione, hanno ritenuto di dovere dare l'assenso all'autorizzazione a procedere, così come richiesta dell'autorità giudiziaria, in particolare dal Collegio per i reati ministeriali. La vicenda è nota: si tratta di un'accusa, ai sensi dell'articolo 323 del codice penale, che viene rivolta all'allora ministro della giustizia Roberto Castelli e ad alcune persone e funzionari privati che avevano concorso, secondo il Collegio per i reati ministeriali, alla concretizzazione di quella fattispecie delittuosa. Mi limiterò a dare alcune indicazioni di carattere giuridico proprio perché sia consentita la valutazione più ampia possibile in questa materia così delicata, perché il Collegio per i reati ministeriali ha ritenuto che la condotta di tutti gli indagati integrasse ed integri, sia sotto il profilo oggettivo sia soggettivo, il reato, così come ipotizzato, di concorso in abuso di ufficio per finalità patrimoniali. Secondo il Collegio per i reati ministeriali era emerso in maniera evidente che nessuno degli incarichi incriminati aveva avuto ad oggetto un'attività di collaborazione nella formazione dell'attività di indirizzo politico del Ministro. Questo va detto perché, a differenza di tanti altri casi precedenti che sono stati giustamente archiviati, anche per quanto riguarda la posizione dell'ex ministro Castelli, questa è una situazione che viene prospettata come diversa e nuova rispetto alle precedenti. Un ulteriore elemento segnalato dal Collegio per i reati ministeriali è che la maggior parte degli incarichi risaliva ad epoca successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 315 del 2001 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 55 dello stesso anno e quindi non sarebbe legittimo fare ricorso e richiamarsi alle previsioni del precedente decreto del Presidente della Repubblica del 1994. Inoltre, andrebbe sottolineato che, in ogni caso, il Ministro non avrebbe effettuato un preventivo accertamento presso le strutture ministeriali, ivi compresi gli uffici di diretta collaborazione, in ordine all'impossibilità di provvedere, con risorse interne proprie del Ministero della giustizia, al raggiungimento del risultato che si proponeva. Continua sempre il Collegio dicendo che nessuno dei consulenti incaricati avrebbe avuto una specifica professionalità in materia e fa in particolare il caso di un dottor Magni, laureato in scienze politiche, definito anche pescivendolo - con rispetto ovviamente per ogni categoria di lavoratori - però ritenuto non adeguato a quello che era l'incarico affidato dal Ministro. Il Collegio per i reati ministeriali segnala inoltre che nessuno dei consulenti nominati avrebbe operato in raccordo con gli uffici preposti, unico interlocutore era risultato essere il Ministro, e inoltre il lavoro dei consulenti medesimi non sarebbe confluito, alla fine, nel patrimonio di conoscenza del dipartimento corrispondente del Ministero. Per quanto riguarda la competenza del dottor Magni, dei viaggi eseguiti ho già detto qualcosa. Conclude le sue osservazioni il Collegio dicendo che risulta approvato anche l'elemento soggettivo, ritenuto necessario per la configurazione della fattispecie delittuosa, di cui all'articolo 323 del codice penale. Di conseguenza, sempre il Collegio ritiene che il comportamento dei membri dei comitati di valutazione sia un comportamento concorsuale rispetto alla fattispecie principale che è stata contestata. Come ha correttamente segnalato nella conclusione del suo intervento il senatore Manzione, si tratta di verificare se ricorra una delle due circostanze esimenti previste all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, cioè in particolare se si è agito per «il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo» oppure se si tratta di un interesse costituzionale particolarmente elevato. elevato. Segnalo che nella relazione del senatore Manzione viene già indicata un'astratta configurabilità illegittima nella condotta degli indagati là dove mette in comparazione il profilo di illegittimità ipoteticamente configurabile rispetto al preminente interesse tutelato. la questione verta su tale valutazione giuridica e, quindi, anche sul comportamento di fatto: se, cioè, è possibile ritenere che l'allora Ministro della giustizia fosse in grado di utilizzare le strutture del Ministero seguendo le indicazioni specifiche della legge, diversamente da quanto ha fatto, oppure se il fatto di agire come Ministro coprisse e possa coprire sempre ed in ogni caso qualsiasi aspetto di illegittimità e di non corrispondenza rispetto a quanto invece previsto dalla normativa specifica.

l'organo di Governo che procedeva esercitasse le proprie funzioni di governo nella riorganizzazione del Ministero, quel comportamento potesse rivestire i profili di illegittimità così come segnalato dal Collegio per i reati ministeriali e che non potesse essere coperto dalla valutazione del preminente interesse pubblico. Il preminente interesse pubblico, infatti, poteva essere tutelato a maggior ragione con il rispetto di tutte le normative (il decreto del Presidente della Repubblica e le circolari presenti in materia). Questa decisione si segnala doverosamente all'Assemblea affinché poi ognuno decida secondo quello che ritiene sia più corretto dal punto di vista normativo.

Il dottor Magni ha fatto il liceo classico e poi si è laureato in scienze politiche. Io l'ho conosciuto nel 1992, quando faceva parte della giunta

tre mandati, a dimostrazione della fiducia che i cittadini nutrivano in lui. Si trattava, pertanto, di una persona che in maniera abbastanza singolare univa un'ottima cultura di base una capacità e ad un'esperienza amministrativa di lungo corso, avendo ricoperto ben tre mandati da sindaco; inoltre, era un imprenditore nel campo della lavorazione del ferro. Siccome è un imprenditore poliedrico, tra le sue varie attività ha iniziato anche un'attività di *import* di grandi partite di pesce (stiamo parlando di interi *container* e di navi intere dall'Africa), che poi rivendeva sui mercati italiani all'ingrosso. Un'attività collaterale, dunque. In base

Questa è la verità dei fatti, questo è il «pescivendolo» che ho incaricato di risolvere i problemi, che ovviamente è stato capace di risolvere. Ci tenevo a dirlo, perché altrimenti magari in

Guardasigilli, che non nominerò, era relativo ad un incarico che riguardava lo studio del processo di attuazione della legge istitutiva del giudice di pace. Era questo un compito che afferiva direttamente al Ministero, sì o no? Risponderanno tutti i colleghi che vorranno trovare una risposta. Molto di più probabilmente di questo che, in modo un po' disadorno, ma forse efficace, il ministro Castelli proponeva ai suoi consulenti; perché per dare una risposta alle cose che diceva il collega Casson bisogna conoscere tutti gli atti e verificare tutte le situazioni. Nel caso di quest'altro Guardasigilli, con un incarico e una consulenza conferiti per un compito che sembra essere corrispondente al ruolo specifico del Ministero, c'è stata l'archiviazione e in questo caso no. Per guardare all'effettività, ho dato conto dei risultati che si sono verificati e che risultano agli atti della Giunta. Per il resto, è evidente che dobbiamo recuperare la capacità di non fermarci alle proposte che ci vengono fatte, a quelle che ci ha fatto il Collegio per i reati ministeriali - e la Giunta non l'ha fatto di non fermarci alle legittime prospettazioni della difesa, e di riuscire a comprendere effettivamente, al di là delle posizioni, che ideologicamente sono tutte legittime, quale sia la reale essenza della vicenda che è al nostro cospetto. Penso di interpretare così la maggioranza effettiva di quella parte della Giunta che ha esaminato gli atti attraverso un percorso lungo e tortuoso, ma proficuo, nella misura in cui ci ha consentito di capire che, al di là delle semplici strumentalizzazioni mediatiche, definire venditore di pesce chi si è laureato alla Cattolica è un'assurdità da non ripetere in quest'Aula; poi ognuno risponde delle cose che vuole affermare. Al di là di questo, però, c'è un contributo effettivo, che alla fine può essere condiviso o meno, ma che rientra in una filosofica filosofica e fisiologica definizione dell'impronta politica che il ministro Castelli ha voluto imprimere al suo Dicastero. In questa logica, politicamente, nella scorsa legislatura ho riempito di critiche il ministro Castelli. Adesso devo solo verificare se la sua impostazione politica coincide con gli atti che ha messo in campo, in una situazione di inagibilità del Ministero della giustizia, che portava il dottor Nebbioso a definirlo disastrato.